*relatore*. Signor Presidente, il testo che è stato approvato dalla Commissione si compone di due articoli e reca disposizioni in materia di tutela dei lavoratori pubblici o privati che segnalino o denuncino reati o altre condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del proprio rapporto di lavoro. Con l'espressione anglosassone *whistleblowing* definita tale pratica - si indica un importante strumento nella lotta alla corruzione che permette di scoprire e, quindi, perseguire illeciti che vengano commessi all'interno delle società. Il *whistleblower*, infatti, è un soggetto che decide spontaneamente di segnalare le violazioni di cui sia a conoscenza, che siano passate, presenti o future. intuizione come tale fenomeno assuma una sempre maggiore rilevanza, soprattutto nello scoprire frodi che altrimenti sarebbero molto difficili da individuare. Il *whistleblowing* è ampiamente conosciuto e regolato negli Stati Uniti - ad esempio - dove, proprio grazie alla collaborazione di di singoli individui, la Security and exchange commission (SEC), un ente governativo che si occupa del controllo dei mercati, ha intrapreso numerose azioni nei confronti di varie compagnie, azioni che hanno portato a sanzioni multimilionarie in capo ai trasgressori. Gli Stati Uniti tutelano da tempo coloro che collaborano alla denuncia di comportamenti fraudolenti o irregolari, permettendone quindi la sanzione. Diverse leggi americane si occupano di regolamentare il *whistleblowing*, prevedendo tutta una serie di vantaggi e garanzie a favore dei singoli *whistleblower*; alcune di queste leggi assumono grande rilevanza anche in Italia e in tutto il mondo, in ragione del loro carattere transnazionale. Non solo in America esistono svariate leggi che regolamentano questo istituto. La sua tutela risulta molto più ampia e dettagliata, prevedendo tutta una serie di vantaggi e garanzie a favore dei singoli *whistleblower*, ed è compresa in una strategia complessiva volta addirittura a incentivare il fenomeno. Il sistema americano prevede - ad esempio - anche misure robuste di premi a favore di coloro che segnalano violazioni e illeciti.

Il disegno di legge in discussione tenta, quindi, di apprestare una prima tutela al fenomeno del *whistleblowing*, senza pretendere di raggiungere subito i risultati di altre legislazioni,

Nello specifico, l'articolo 1 modifica l'attuale disciplina riferita ai lavoratori pubblici di cui all'articolo 54-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001, mentre l'articolo 2 concerne i lavoratori del settore privato. La riforma, pur confermando il principio di tutela già in vigore, in base al quale l'autore della segnalazione o della denuncia non può essere sottoposto a misure aventi effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, presenta una serie di elementi di novità. L'ambito di applicazione della disciplina è esteso ai lavoratori pubblici diversi dai lavoratori dipendenti (collaboratori o consulenti), nonché ai lavoratori, collaboratori e consulenti degli enti pubblici economici, a quelli degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, ai lavoratori e ai collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzino opere in favore dell'amministrazione pubblica. Le disposizioni previste si applicano alle segnalazioni effettuate nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione. Riguardo ai possibili soggetti destinatari della segnalazione, la novella sostituisce il riferimento al superiore gerarchico con quello al responsabile della prevenzione della corruzione: figura presente in ogni pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012. Resta ferma l'ipotesi di segnalazione all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) o di denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile. In merito al principio di tutela, si prevede che l'adozione di misure ritenute ritorsive sia comunicata in ogni caso all'ANAC, da parte dell'interessato o delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, informi il Dipartimento della funzione pubblica o gli altri organismi di garanzia per le determinazioni di competenza. A tale proposito, si ricorda che la norma vigente prevede, invece, che l'interessato o i sindacati segnalino le misure ritenute discriminatorie al Dipartimento della funzione pubblica. Si introduce, per il caso di adozione di una misura discriminatoria, una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro, a carico del responsabile che abbia adottato la misura, fermi restando gli altri profili di responsabilità Si introduce l'inversione dell'onere della prova a carico del datore di lavoro, il quale dovrà dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, siano motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa, stessa, confermando la nullità degli atti discriminatori o ritorsivi adottati dal datore di lavoro nei confronti del lavoratore. E, qualora ne venga accertato l'illegittimo licenziamento, si dispone il reintegro nel posto di lavoro, anche con ordinanza ingiuntiva del tribunale, oltre al risarcimento per eventuali danni morali, economici o di carriera subiti nonché al rimborso delle spese legali sostenute. La sussistenza di una misura discriminatoria è accertata dall'ANAC, che è altresì competente a irrogare la relativa sanzione. Si modifica anche la tutela della riservatezza circa l'identità dell'autore della segnalazione, limitando la vigente deroga al principio di riservatezza al caso in cui la conoscenza dell'identità sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, purché la contestazione sia fondata, anche solo parzialmente, sulla segnalazione e solo in presenza di consenso da parte dell'interessato. Si conferma, invece, che alle segnalazioni in oggetto non si applica la disciplina sul diritto di accesso agli atti di cui alla legge n. 241 del 1990. È affidata all'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, la predisposizione di linee guida per la presentazione e la gestione delle segnalazioni che garantiscano la riservatezza del dipendente segnalante.

il mancato svolgimento di attività di verifica delle segnalazioni ricevute da parte del responsabile, applicando a quest'ultimo una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Medesima sanzione è prevista nei casi di assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni, ovvero nei casi di adozione di procedure non conformi a quelle predisposte dall'ANAC. Come è facilmente intuibile, la scelta di aumentare le sanzioni nei casi di assenza delle procedure per la segnalazione e nei casi di mancato riscontro delle segnalazioni ricevute è dovuta alla volontà di prevenire condotte omissive che avrebbero effetti diretti sulla funzionalità e sull'efficacia della segnalazione stessa. L'applicazione delle tutele non è garantita nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la medesima segnalazione, ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. L'articolo 2 del disegno di legge di legge estende al settore privato la tutela del dipendente o collaboratore che segnali illeciti, attraverso modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 231 del 2001. In particolare, è integrata la disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti privati derivante da reati. La disciplina concerne gli enti, società e associazioni (anche prive di personalità giuridica) privati, nonché gli enti pubblici economici. In base a questa normativa, essi sono responsabili per i reati commessi da determinati soggetti nell'interesse o a vantaggio dell'ente. quest'ultimo è esclusa qualora ricorrano alcune condizioni, tra cui l'adozione e l'attuazione di modelli di organizzazione e gestione aventi determinati requisiti. Le novelle all'articolo 6 del decreto legislativo n. 231 del 2001 integrano i requisiti stabiliti per i suddetti modelli. Nello specifico, essi devono contemplare, a carico di coloro che a qualsiasi titolo dirigano o collaborino con l'ente, l'obbligo di presentare segnalazioni circostanziate di illeciti o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Si prevedono canali alternativi di segnalazione, di cui almeno uno idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante, nonché misure idonee a tutelare l'identità del segnalante e le relative sanzioni nei confronti di chi violi le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettui, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelino infondate. È previsto il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati alla segnalazione. Si specifica, inoltre, che l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuino le segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo. Infine, anche per il settore pubblico, si sancisce la nullità dei licenziamenti o di altre misure ritorsive o discriminatorie, adottati nei confronti del segnalante, ivi compreso il mutamento di mansioni, e si pone a carico del datore di lavoro l'onere della prova che le misure organizzative adottate successivamente alla segnalazione siano fondate

premettendo che noi riteniamo che la corruzione e la violazione della legge nell'ambito della pubblica amministrazione a danno dell'Erario pubblico siano reati gravi da perseguire con efficacia e determinazione.

Con le norme approvate dall'altro ramo del Parlamento - e meno male che l'altra Camera non sia l'unico ramo del Parlamento, come lo sarebbe stato se fosse passato il *referendum* dello scorso 4 dicembre - è sufficiente è sufficiente una segnalazione, ad esempio, all'Autorità nazionale anticorruzione per garantire il posto, per un tempo indeterminato, a chiunque abbia rapporti economici con le pubbliche amministrazioni. Poiché il provvedimento ha il nobile proposito di proteggere coloro che forniscono elementi utili a individuare irregolarità nell'ambito della pubblica amministrazione

tanto meno licenziate o essere addirittura oggetto di misure organizzative aventi effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinate dalla segnalazione.

che venga accorpato a un altro e, dunque, verosimilmente venga spostato anche dal punto di vista geografico con evidente disagio. Una persona che ha il lavoro vicino a casa non è contento, di essere

la medesima disciplina si applica anche ai collaboratori e ai consulenti con qualsivoglia tipologia di contratto e incarico, nonché ai lavoratori e collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni e servizi che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica? Può accadere che una persona - per esempio - di un'impresa di pulizie, assunta temporaneamente

la quale lavora. Non si capisce neppure come si possa applicare. Vuol dire che questo lavoratore deve essere stabilizzato fintantoché il giudice non stabilirà l'infondatezza della sua segnalazione? Qui abbiamo veramente una grave

sono stati molto pochi e francamente - a mio parere - non decisivi, nonostante la buona volontà del relatore e dei componenti della Commissione competente. Ecco perché proponiamo di non procedere con l'esame del provvedimento, la cui efficacia - temo - si manifesta in particolare nel settore privato. Si corre il rischio che non ci siano più

più scarse. Pertanto, perde il lavoro. È remotissima la possibilità di segnalazioni infondate o strumentali. Invece, abbiamo una sorta di stabilizzazione. Mentre con i nuovi contratti di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, introdotti dal *jobs act*, in pratica non

ogni passo può essere soggetto a delazione o calunnia strumentate a stabilizzare il proprio posto di lavoro, addirittura di un collaboratore temporaneo di una ditta esterna, non ci sarà alcun dirigente

Altro che tutela dei lavoratori. Rischiamo di far sparire centinaia di migliaia di posti di lavoro in nome di un principio di pangiustizialismo che, invece, dovrebbe orientarsi su un aspetto molto semplice: quando c'è il reato, deve essere punito e chi lo segnala deve essere tutelato. Questa dovrebbe essere la norma, molto semplice, che in grandissima parte già esiste; qualcosa probabilmente poteva essere

vorrei far presente al collega Malan che non è vero il presupposto del suo intervento. La norma dice che sono vietati gli atti di ritorsione o discriminatori motivati o discriminatori motivati direttamente o indirettamente dalla segnalazione. Questa non è altro che la specificazione di un principio generale del nostro ordinamento, contenuto già nell'articolo 15 dello statuto dei lavoratori,

rappresaglia contro un comportamento lecito del dipendente o del collaboratore (perché il principio di non discriminazione non è limitato all'ambito del diritto del lavoro subordinato). Dunque la norma che il collega Malan denuncia non è altro che una specificazione, in riferimento a questa materia, di un principio che già esiste nel nostro ordinamento e che già potrebbe applicarsi nel caso specifico anche se questa disposizione non venisse non venisse introdotta da questo disegno di legge. Per altro verso, invito i colleghi a considerare la situazione di grave imbarazzo in cui si trova il dipendente, di un'amministrazione pubblica o di un'impresa privata, che, per ragione dello svolgimento dei propri compiti, venga a conoscenza di una qualche notizia che potrebbe essere la punta dell'*iceberg* di una pratica illecita, di una malversazione, di un episodio di corruzione, ma potrebbe anche non esserlo. Il lavoratore, il dipendente, l'impiegato oggi non è in grado di in alcun modo. Infatti, se per ipotesi la notizia fosse coperta da segreto aziendale, d'ufficio o professionale (articolo 622 del codice penale) e e si rivelasse, poi, non corrispondente a un episodio di malversazione, indipendentemente dalla sua buona o cattiva fede, il dipendente potrebbe essere in futuro perseguito per violazione, appunto, dell'obbligo di segreto. Il disegno di legge offre al dipendente che si trovi in questa scomoda e difficile situazione lo strumento appropriato, cioè il canale riservato attraverso cui comunicare la notizia, senza che la rivelazione possa provocare danno al soggetto attivo dell'obbligo di segreto professionale, aziendale o d'ufficio, a un organo che fungerà da filtro e saprà distinguere ciò che merita di essere approfondito e ciò che invece non ha rilievo; e chi

In questo vedo soltanto il perfezionamento di una disciplina generale del segreto professionale, aziendale o d'ufficio, che oggi, su questo tema, lascia una zona di incertezza, una zona grigia, nella quale troppo spesso l'indeterminatezza l'indeterminatezza della regola di comportamento favorisce un silenzio che nasce da una malintesa prudenza, dalla paura di possibili conseguenze. Il disegno di legge mira a favorire il comportamento corretto del cittadino, del dipendente, dell'impiegato pubblico che vuole fare la propria parte anche senza sapere fino in fondo quali sono le conseguenze della sua rivelazione, ma con la preoccupazione - per recare danno laddove la notizia possa portare un danno ingiusto a qualcuno. Signor Presidente, colleghi, viviamo per il momento in un Paese democratico, in Stato di diritto e credo che dovremmo cercare di evitare di incamminarci lungo la china dello Stato di polizia.

un possibile non rispetto delle norme penali sono già previste garanzie e, ovviamente, le procedure che possono consentire al cittadino leale, che collabora con lo Stato, la segnalazione del fatto e le tutele conseguenti. Non possiamo accettare di creare una normativa

di attività che devono essere necessariamente puntuali e approfondite, perché altrimenti potrebbero portare a gravi lesioni dei diritti dei cittadini sospettati.

accettare l'idea che i cittadini onesti sono in grado di svolgere la propria funzione senza avere protezioni particolari che potrebbero indurre invece cittadini disonesti a imboccare la strada del regolamento di conti, della vendetta e di tante altre situazioni che, purtroppo, possono coinvolgere l'essere umano. Un Paese democratico, un Paese che in cui lo Stato di diritto è saldo non ha bisogno di norme di questo genere.

Dico «batterci» perché credo che, a questo punto, siamo arrivati a un nodo cruciale del discorso generale che in questa legislatura è stato sfiorato più volte, toccato, modificato, peggiorato,

un sicofante, un delatore. Risparmiamoci tutta la tiritera sul nome, la mancata traduzione e tutte le difficoltà; fatto sta che in questo Paese

e Buemi si annidi un grosso equivoco e cioè confondere la segnalazione con la denuncia. Quando parliamo di segnalazione parliamo di elementi,

un gesto profondamente immorale, che è andato a danno della corretta fiscalità di molti Paesi, tra i quali anche l'Italia, cui ha sottratto risorse. Rimanendo sul punto delle risorse e a quello che il senatore Malan non dice, che il senatore Maran ha solo accennato quando ha parlato di ciò che accade negli Stati Uniti, forse varrebbe la pena di aggiungere che negli Stati Uniti è proprio il meccanismo del *whistleblowing* che ha permesso di recuperare

Questo è un comportamento che coinvolge soprattutto i giovani, che arrivano in un luogo di lavoro credendo in un mondo pulito

di essere oggetto di ritorsioni. Anche questo è vero: non possiamo nasconderci dietro ai discorsi paludati di chi non ammette che la realtà è diversa. Senatore Buemi, la realtà è diversa: oggi

rivolgersi e deve tacere per non perdere il lavoro e le sicurezze familiari. Credo davvero che chi oggi pensa che questo sia un

riusciti ad affrontare in modo serio la corruzione. Si tratta di un'opera di prevenzione per la quale dobbiamo invocare la responsabilità di ogni singolo che compone questo popolo, ma dobbiamo anche metterlo nelle condizioni di essere sicuro di non pregiudicare

Esistono o non esistono nel nostro ordinamento garanzie e procedure di tutela per chi segnala reati o irregolarità di cui sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio rapporto di lavoro? Secondo questa proposta, non ci sarebbero o sarebbero insufficienti e lacunose. Se così fosse, il nostro ordinamento - ha ragione il collega Buemi - non sarebbe affatto quello di uno Stato di diritto la nostra organizzazione costituzionale presenterebbe lacune e incertezze di proporzioni enormi. Io non penso che sia così; ho invece la netta sensazione che, attraverso queste misure, abbandoniamo un terreno di garanzie e procedure di tutela per inoltrarci in quello scivolosissimo e, sotto certi aspetti, ripugnante delle protezioni "particolari". Metto la parola particolari tra virgolette, ritenendo che non sia questo il momento per inoltrarci in profili di legislazione comparata tra gli Stati Uniti d'America e il nostro Paese, perché allora il discorso deve investire non solo

di fissare una distinzione tra semplici segnalazioni e vere e proprie denunce,

all'epoca delle cosiddette mani pulite ci fu un imprenditore molto brillante (mi pare che fosse allora amministratore delegato della FIAT), il quale si recò dai magistrati del *pool* di Milano

Fu quello un momento molto brutto e ripugnante della nostra storia nazionale. Vada poi, se ci riesce, in sede di ricostruzione storica, magari aiutata dall'immancabile dottor senatore onorevole Di Pietro, in trasmissioni televisive a ribadire che una cosa sono le semplici segnalazioni e una cosa sono le denunce vere e proprie. Prendiamo ad esempio l'articolo 2 del testo l'articolo 2 del testo proposto dalla Commissione. Mi dispiace che ciò sia sfuggito a un collega attentissimo su queste questioni, come il senatore Ichino. Si parla di «uno o più canali che consentano ai soggetti indicati (…), a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte». A norme di questo genere mi si dice che si era già pensato nel passaggio tra la Russia e l'Unione Sovietica.

che quest'Assemblea non si ponga, e che il relatore ha in qualche modo bypassato: come è possibile che questo testo arrivi in Aula senza essere passato

a giudizio del nostro Gruppo sono molteplici. Di qui, il nostro voto favorevole e la nostra gratitudine al collega Malan per l'attenzione che ha dato a questo testo. *(Applausi Presidente, colleghi, non posso credere che qualcuno qui dentro ritenga la corruzione qualcosa di diverso da una serpe che va schiacciata. Abbiamo a che fare con il pericolo, con il nemico più grande e più grave della pubblica amministrazione, dello Stato italiano e del popolo italiano nel suo complesso. Non posso pensare che qui si ritenga

quando sappiamo benissimo che chi denuncia riceve minacce. Lo abbiamo visto finanche nel mondo dell'università: guai a te se ti presenti al concorso, perché finisce la tua carriera! dunque a queste persone che noi dobbiamo dare tutela, agli eroi che mettono la faccia per l'interesse di tutti. Non posso pensare che si ribalti, con un teorema artificioso, il ruolo di chi deve essere tutelato con quello di chi deve essere combattuto. Quando si schiaccia una serpe senz'altro questa si contorce: cerchiamo di fare in modo che sia la serpe a contorcersi e non qualcuno qui dentro a sollevare equilibrismi, artifizi, cavilli per negare l'evidenza. Abbiamo un pilastro della lotta anticorruzione: emergere il malaffare. Un altro pilastro è che si celebrino con certezza i processi. Un altro pilastro ancora è che si comminino pene efficaci. Il Movimento 5 Stelle ha presentato proposte importanti su tutti e tre i fronti: la riforma della prescrizione e il DASPO ai politici corrotti. Ma qui dobbiamo agire sul precursore di queste possibilità, cioè sul fatto che ai cittadini sia data la possibilità di conoscere ciò che accade. E non spetta a chi segnala certificare se si tratta di un fatto con rilevanza penale o meno, spetta alla magistratura ed è nel rispetto di queste competenze che il cittadino deve essere messo nelle condizioni di dire quello che sa, rimettendo ad altri il compito di valutare. viene vessato, viene messo di fronte a una museruola preventiva e non ha le tutele dopo che gli spettano di diritto, come avviene in altri Paesi, allora noi blocchiamo sul nascere tutta questa catena di interventi contro la corruzione. Non solo, allora, rimaniamo un Paese che è indietro rispetto ad altri su una normativa virtuosa, ma questo Paese è destinato ad arretrare. Ora andremo a votare su questa pregiudiziale e noi la respingeremo con decisione e si vedrà, da questo, anche chi ha cuore o meno il bene del Paese.

che è mera traduzione, dal *common law* al nostro ordinamento legislativo, di una disciplina priva di certezze, soprattutto per la continuità dell'amministrazione pubblica.

Se fossimo stati in Commissione giustizia avrei chiesto cosa volesse dire la denuncia di una violazione del modello di organizzazione e gestione dell'ente: perché, un dipendente privato può segnalare una violazione della gestione dell'ente, scavalcando anche il sindacato? Ma di cosa stiamo parlando? Perché non abbiamo avuto l'occasione in Commissione giustizia di esaminare un provvedimento, che io vedo adesso per la prima volta? Come membro della Commissione giustizia non ho avuto la possibilità, che il Regolamento del Senato mi garantisce, di poter approfondire un argomento così importante. Altro che lezioni di legalità! Cominciamo a rispettare qua la legalità.

Comunque, adesso c'è la possibilità di fare tutto.

«Che fai, ricorso? Però così ti giochi la carriera». Comunque si trova in Aula, senatore Giovanardi. Adesso procediamo con la discussione generale, così come ho disposto. Prego, senatrice Montevecchi.

«Che fai, ricorso? Però così ti giochi la carriera». Questo sembra abbia detto il professor Pasquale Russo a Philip Laroma il 21 marzo 2013 in una conversazione telefonica. Questo accadeva all'interno di un ateneo, quello di Firenze, dove pare ci fosse un professore che tentava di garantire ad un proprio pupillo un posto come docente nel futuro concorso. Nonostante nel 2012 sia stato introdotto, con la legge Severino, l'istituto del *whistleblowing* e quindi sia stata riconosciuta la figura del *whistleblower*, in realtà,

prima dell'approdo del disegno di legge in quest'Aula ancora si doveva mettere mano ad un miglioramento delle tutele previste per chi ha il coraggio di denunciare queste attività illecite all'interno degli atenei. Tanto che quando scoppia il caso, che investe anche atenei di altre Regioni italiane, tra cui l'ateneo della mia città, Bologna, gli studenti intervistati, seppure indignati, si sono dimostrati rassegnati, proprio perché ormai questi fatti dilagano, sono normale amministrazione. Questo costume porta con sé un carico pesante, perché significa togliere ai nostri giovani ogni ogni prospettiva, significa togliere ai nostri giovani il futuro, la possibilità di sperare di poter fare carriera all'interno dei nostri atenei sulla base del proprio merito e non su meccanismi di clientela o di filiazione

il futuro dei nostri giovani, oltre che riconoscere il merito delle persone che con coraggio mettono in discussione sé stessi, la propria famiglia, il proprio posto di lavoro, quindi la propria stabilità, pur

non va. Mi auguro che questo disegno di legge, che porta la firma di diversi nostri colleghi, possa finire il proprio *iter* in questa legislatura e spero davvero che non si faccia alcunché per affossarlo, perché il tentativo di affossare questo disegno di legge, lo ribadisco, sarebbe il tentativo di togliere a tante persone la tutela e il coraggio per poter denunciare, che stanno alla base di una bonifica di certi ambienti, come quello universitario, che sono fondamentali non solo per la formazione personale dei nostri giovani, ma anche per il futuro stesso di questo Paese, perché da quelle aule escono i nostri migliori cervelli e hanno diritto a fare una carriera dignitosa basata sul merito e dare gloria a questo nostro Paese. colleghi, finalmente arriva in prossimità dell'approvazione un testo di legge che è fondamentale per combattere un male endemico del nostro Paese, nostro Paese, quello di una corruzione diffusa che ha ulcerato i tessuti più molli della pubblica amministrazione venendo anche a danneggiare gangli che con la pubblica amministrazione entravano in rapporto, cioè i gangli dell'economia privata, perché la corruzione, e questo lo sappiamo, non è più un problema della cosiddetta PA, ma è un problema di tutti quei soggetti che, entrando in rapporto con la PA, vengono ad essere infettati dalle malattie della pubblica amministrazione stessa. Ora, io ricordo a me stesso che sarebbe il caso di ascoltare chi combatte da tanto, tanto tempo questi fenomeni corruttivi che sono, come diceva poc'anzi la mia collega Montevecchi, quei fenomeni che fanno rassegnare coloro che non debbono rassegnarsi. Benissimo, da tempo tanti magistrati ancora in attività scrivono fornendo dei suggerimenti in base alle esperienze che loro stessi hanno vissuto e uno dei magistrati che mi sembra più degli altri abbia lavorato a questi problemi indicando soluzioni è, per uno di quelli che non stanno tanto simpatici né alla mia sinistra, né alla mia destra, e cioè Piercamillo Davigo. *(Brusio)*. Sento commenti. Sì, forse c'è qualcuno cui duole, che soffre nel sentire certi nomi, nomi che a me ricordano quanto sia doveroso combattere per la giustizia. Quando ricordo gli insegnamenti e le riflessioni molto, molto amare di Piercamillo Davigo ma anche di altri, non soltanto quelli che facevano parte del *pool* di mani pulite ma anche di quelli che in tante procure, molto meno famose, hanno avuto difficoltà a combattere fenomeni di corruzione, io ricordo che il problema è di natura culturale perché, come ribadiva la senatrice Mussini, qui la segnalazione viene considerato da tanti, da troppi, come delazione: che fai, parli? Che fai, denunci? Che fai, segnali? Allora, noi dobbiamo metterci in testa una cosa: la corruzione è un fenomeno endemico e massivo ed è possibile quando gode di coperture tali per cui tutti quanti volgono lo sguardo altrove. Una vicenda emblematica proprio di questa perniciosità e di questa endemicità del fenomeno è quella di tale Andrea Franzoso, che ha denunciato, all'interno di Ferrovie Nord, qualcosa che non andava e che poi ha pagato caro ed amaro questo suo esser ligio nei confronti della giustizia. Non può essere che chi denuncia e chi segnala venga lasciato solo, dovendosi magari anche sobbarcare oneri legali,

Questo è stato capito da ordinamenti giuridici che non lasciano soli i cittadini che denunciano, piuttosto li affiancano e li tutelano. Anche perché, caro Presidente, lei insegna che chi effettua una segnalazione non corre alcun problema, perché una segnalazione non è una denuncia, ma chi effettua una denuncia, che poi si dovesse ravvisare falsa e infondata, commette lui stesso un reato e pertanto deve essere particolarmente

L'Italia è il Paese dell'omertà, è il Paese in cui è normale che anche in quest'Aula si violi il Regolamento, votando, per esempio, per i colleghi assenti, senza che tutto questo crei problemi e dia scandalo. Se vogliamo ripristinare una cultura della giustizia che sia effettiva e solida, se vogliamo, per esempio, come ribadiva il senatore Endrizzi, parlare di certezza del diritto, dobbiamo fare in modo che le regole, anche quelle inadeguate e approssimative (perché le regole sono figlie di noi essere umani e quindi sovente possono essere sovente possono essere sbagliate), vadano comunque rispettate, fermo restando che chi sposa la filosofia della disobbedienza civile può anche acconsentire di andare contro la regola accettando, parimenti, di andare incontro alla sanzione prevista per chi infrange la regola. E allora ben venga, seppur a conclusione di legislatura, un testo, magari non perfetto e in alcuni casi da affinare, che finalmente pone al centro non tanto chi segnala, quanto piuttosto la doverosità per il cittadino e per il lavoratore di far emergere situazioni anomale, irregolari mi lasci usare questo termine - bastarde. Questo Paese è stanco di dover ricordare eroi, che altrove non sono tali perché non sono soli, ma sono accompagnati da frotte, da stuoli di cittadini che hanno coscienza di cosa sia dovere fare e segnalare - perché il termine *whistleblower* questo significa: il segnalatore - non è affatto essere delatori. Nell'antica Atene lo psicofante era un fetente e un traditore e magari in alcune zone del nostro Paese, ove vige una cultura criminale - e lei queste zone le conosce meglio del sottoscritto - sa che non parlare

a Paesi che vogliono combattere la corruzione. Se tutti, da destra a sinistra, capissimo la necessità di promuovere certe battaglie, questo sarebbe un Paese in cui il Movimento 5 Stelle non avrebbe ragion di esistere. Ma se questo è, è perché per troppi decenni questa legislazione è stata annunciata, magari anche con un *tweet*, e poi negata. Portiamo dunque a termine il lavoro e, lasciando stare le polemiche d'Aula, cerchiamo un pochino di concludere un onere che ci darà molti onori, perché permettere ai cittadini di far giustizia non è affatto una cosa sciocca e neanche banale.

legiferi sotto forma di repressione, ma non in forma preventiva. suonato come campanello d'allarme, ma che probabilmente non abbiamo avuto la capacità di interpretare nel giusto modo. Con il termine anglosassone *whistleblowing* - oramai siamo pieni di

la violazione di una legge, collaborando così alla punizione dei comportamenti dei trasgressori. Esso viene considerato uno strumento di particolare aiuto alla lotta alla corruzione, che, come si è già detto, probabilmente non ha fine in questo Paese. Questo disegno di legge prevede innanzitutto una modifica dell'articolo 54-*bis* del decreto legislativo 165 del 2001, che già tutela il pubblico dipendente che denuncia condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro. Denunciare forse è una parola forte, ma che viene esplicitata come segnalazione in buona fede quando il soggetto sia mosso dalla ragionevole convinzione che la condotta illecita si stia verificando. Si cerca di proporre un rafforzamento dell'anonimato del singolo e di tutelare la riservatezza dell'identità del segnalatore. Vengono previste sanzioni amministrative pecuniarie nel caso in cui l'ente ricorra a trattamenti discriminatori nei confronti del dipendente denunciante. La maggiore novità di questo provvedimento è la parte che riguarda la tutela del dipendente o collaboratore che segnala condotte illecite nel settore privato. Qui la modifica viene fatta al decreto legislativo n. 231 del 2001. In particolare, è previsto il dovere da parte di chi riveste funzioni di direzione dell'ente, nonché di chi collabora a qualsiasi titolo con l'ente stesso, di presentare segnalazioni di illeciti che ritengono si siano verificati. La norma prevede il divieto delle misure discriminatorie nei confronti di questi *whistleblower*, la cui violazione comporta una denuncia all'Ispettorato del lavoro, del lavoro, ed è chiaramente nullo il licenziamento e i mutamenti di mansioni ritenuti ritorsivi nei confronti del segnalatore. Questi due articoli cercano di dare seguito applicativo alla cosiddetta legge Severino, che pure aveva contemplato l'articolo 1, comma 51, che prevede l'obbligo per ogni pubblica amministrazione di dover tutelare il dipendente che segnali illeciti all'interno dell'ambiente di lavoro. La legge Severino enunciava un principio, ma non creava gli strumenti utili alla sua concretizzazione. L'Autorità nazionale anticorruzione sta cercando di dare concretezza alle previsioni già contemplate, ma palesa anche i limiti dei poteri nel gestire i casi di discriminazione, arrivando a sostenere che essa può mettere in campo un'attività per il futuro e non per il passato. Vediamo qual è il senso di questo disegno

Non l'ho trovato perché sia nel testo unico del pubblico impiego che nel diritto del lavoro i dipendenti che denunciano reati non possono essere né sanzionati, né licenziati, né tantomeno mobbizzati e, se ciò avvenisse, chi lo fa, correttamente, viene punito per il reato. Chi lo fa commette, a sua volta, chiaramente degli illeciti disciplinari. A mio modesto avviso, credo ci siano già tutte le norme per punire i reati di abusi sia nel settore pubblico che in quello privato.

Lega Nord alla Camera, lo fate per andare sui giornali domani mattina perché qualcuno di voi possa apporvi la propria firma. Con questo provvedimento si crea un potere forte e uno squilibrio tra chi accusa e chi si trova costretto a difendersi, squilibrio troppo a favore del dipendente o di alcuni dipendenti. Già solo questo dimostra la poca

Non si può perseguire questo nobilissimo obiettivo con gli incentivi come se stessimo parlando di pannelli solari. Signor Presidente, se ci fosse uno di questi

Signor Presidente, mi consenta una precisazione: nell'antica Grecia c'era il sicofante o delatore prezzolato e non lo psicofante, che forse è un neologismo e una figura più adatta ai nostri tempi. Detto questo, vorrei fare alcune considerazioni il più possibile oggettive. In Italia già oggi vige il principio per cui il pubblico dipendente che venga a conoscenza sul posto di lavoro, nell'esercizio delle sue funzioni, di un reato ha l'obbligo di denunciarlo. Un testo di legge già in vigore stabilisce che, fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, il pubblico dipendente che denuncia condotte illecite, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto a una misura discriminatoria. Questa è la legge Severino, che il Parlamento ha approvato quattro anni fa. Il primo problema che ci pone il disegno di legge che stiamo esaminando oggi è quello della sua effettiva necessità. Stiamo facendo un doppione? La domanda mi sembra lecita perché si potrebbe fare riferimento, oltre che alla legge Severino, anche al decreto legislativo n. 165 del 2001 per quanto riguarda la pubblica amministrazione, al decreto legislativo n. 231 del 2001 per quanto riguarda l'impresa privata

pubblico, sia nel settore privato. Secondo punto: si è introdotto in questa proposta di legge il principio dell'obbligatorietà della denuncia anche nei confronti del cittadino privato. Il nostro ordinamento non prevede che il privato cittadino sia obbligato a denunciare i reati di cui sia venuto a conoscenza. Se assisto a un furto non ho il dovere di andare dai carabinieri, tranne nel caso in cui si tratti di reati contro la personalità dello Stato. Nel caso del pubblico impiegato non c'è invece delazione, perché è lo Stato stesso che si difende ed esercita un diritto-dovere nel proprio interesse. Il privato, invece, non ha questo diritto dovere e quando si arriverà all'applicazione concreta di questo provvedimento si porrà il problema della sua costituzionalità. Ma c'è un altro problema in materia di applicabilità di queste norme nell'ambito delle strutture economiche private. È chiaro che nelle aziende molto piccole una norma di questo genere aggiunge una serie di obblighi che comportano oneri non indifferenti sul piano economico, per cui sarebbe opportuno almeno limitarne l'applicabilità alle aziende maggiori o a quelle che utilizzano capitali di rischio. Più in generale, è difficile accettare che per chi denuncia venga prevista una sorta di premialità, mentre c'è poco o nulla a garanzia del denunciato. Se denunciare è un dovere, perché chi lo fa deve essere premiato? E per chi è accusato, se venisse poi prosciolto,

tutelare i denunciati. Questo disegno di legge nasce sull'illusione che, incentivando la delazione, si possa migliorare l'etica pubblica. Infine, la questione ANAC. L'ANAC è di fatto un giudice collaterale a tutti gli altri giudici. Oggi non contano più i TAR, non conta più il giudice penale; l'ANAC è capace, con un suo provvedimento, di giudicare oltre i TAR, oltre il Consiglio di Stato, oltre il giudice penale. Anche su questo dovremmo fare una profonda riflessione in un sistema che è fondato costituzionalmente su organi di giurisdizione precodificati e preindicati. *(Applausi dei